Il 1° marzo l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento. Il relatore facente funzione,

giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 486, a prima firma della senatrice Murelli, che ringrazio per la lodevole iniziativa, approvato all'unanimità dalla 7a Commissione permanente lo scorso 7 marzo. Il provvedimento mira a riconoscere il Teatro Regio di Parma quale monumento nazionale. Nel corso dell'esame in sede redigente, la Commissione non ha apportato modifiche al testo dei proponenti. Il disegno di legge in esame recepisce i contenuti di analoga iniziativa legislativa, a prima firma della senatrice Saponara, che, nella scorsa legislatura, venne approvata dal Senato in prima lettura e trasmessa alla Camera. Quest'ultima non ne poté tuttavia concludere l'esame, per via della conclusione anticipata della legislatura. Il provvedimento si compone di due articoli: l'articolo 1, ai sensi del quale, come detto, il Teatro Regio di Parma è dichiarato monumento nazionale nel testo originario, e l'articolo 2, che dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento in esame. Il Teatro Regio, in origine Teatro Ducale, venne edificato per volontà della duchessa Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, moglie di Napoleone, che resse il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dal 1816 al 1847. La duchessa, amante della musica e del canto, nel prendere atto che il vecchio Teatro Ducale, fondato nel 1689, era inadeguato alle esigenze della città, promosse la realizzazione di un nuovo edificio più moderno. Il Teatro, in stile neoclassico, in origine era destinato ad accogliere forme diversificate di spettacolo, quali l'opera, la danza e la recitazione di poesie, sino ad includere attività assimilabili agli attuali spettacoli circensi. Sin dalla sua inaugurazione, il Teatro Regio di Parma è testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante l'Ottocento e il Novecento, dalla fine dell'epoca legata al nome di Rossini alla supremazia del repertorio verdiano, dall'apertura alle esperienze francesi e tedesche all'opera italiana con Mascagni, Leoncavallo e Puccini. Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro, di cui all'articolo 1, è volta a riconoscere, direttamente con norma legislativa, l'indiscutibile rilievo culturale del medesimo e l'attività artistica che in esso si è svolta, e continua a svolgersi, sin dalla sua inaugurazione. La norma appare peraltro in linea con la dichiarazione di monumento nazionale della casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto, riconosciuta con la legge 3 febbraio 1901, n. 26. Entrambi questi luoghi, infatti, hanno avuto un significato rilevante nella vita del maestro. La dichiarazione di monumento nazionale, alla luce di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, costituisce un riconoscimento di quei beni culturali che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico

si pone in linea con altri interventi di rango primario, fra cui è possibile ricordare la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica palladiana di Vicenza, la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazioni di monumento nazionale della casa museo Gramsci a Ghilarza, la legge n. 213 del 2017 che ha dichiarato monumento nazionale la casa museo Matteotti a Fratta Polesine e la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto Ponte vecchio di Bassano.

Riconoscere oggi il Teatro Regio come monumento nazionale, di valore storico, in un certo senso completa il percorso fatto in questi due anni e sottolinea ancora più la centralità della cultura a Parma. Parma, una città che in questi giorni sta avendo grandi soddisfazioni per quanto riguarda la fiera, con l'accordo fatto anche con la fiera di Milano, sempre più *food valley* e sempre più al centro di interessi economici, diventa capitale culturale ancora più forte. Il Teatro Regio, Il Teatro Regio, famoso per le opere verdiane, non è un teatro lirico-sinfonico, ma è un teatro di tradizione. Per questo chiedo ancora una volta al Governo che, nonostante questo *handicap*, non venga escluso dai festeggiamenti per i duecentodieci anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. Sarebbe uno scippo ingiustificabile

L'orchestra Toscanini è fatta di giovani professionisti, molto bravi e preparati, che meritano il rispetto e il giusto riconoscimento del mondo culturale nazionale e regionale.

nei banchi della maggioranza l'ha riproposto favorendo un percorso veloce, che da oggi darà la possibilità al Teatro Regio di Parma di essere un monumento storico.

il fruitore, il cittadino, non è solo spettatore passivo, perché insieme all'artista vive un momento irripetibile, magico, in un luogo unico, con una tensione emotiva. Il teatro è, quindi, una forma d'arte riproducibile nell'epoca della riproducibilità. Il Teatro Regio di Parma è un centro nevralgico della cultura musicale italiana, da cui sono passati gli artisti più importanti. Nel palco hanno manifestato la grande tradizione operistica italiana artisti come Luciano Pavarotti, Carreras, Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Maria Callas e Renata Tebaldi. È anche un luogo straordinario per le caratteristiche architettoniche di impronta neoclassica e artistiche, con la camera acustica decorata, dipinta a tempera, e con sale affrescate che conservano ancora le arie di Verdi e di Bellini; ma lo è soprattutto per il vissuto sociale che ha caratterizzato negli ultimi due secoli quel Teatro. La dichiarazione di monumento nazionale, a mio avviso, deve considerare non il singolo edificio, non il luogo in sé nella sua esteriorità, ma ciò che quel luogo ha rappresentato, ciò che ha contenuto, cioè le dimensioni che appartenevano a persone, uomini e donne, la memoria di vita. Il Teatro Regio di Parma rappresenta una visione culturale più complessiva: un Teatro che non si ferma dentro le mura, ma che esce e va nella città a incontrare interi quartieri di gente per dialogare con loro, con le persone anche più svantaggiate. Una visione di sviluppo di una città che promuove eventi di coesione, di legame sociale collettivo senza riferimenti ossessivi alla pura razionalità utilitaristica, per rafforzare nei cittadini la voglia di vivere, quell'istinto ricreativo e vitale che è in ognuno di noi, che ci salva dalla solitudine e dalla depressione, che abbiamo visto, anche in questa Aula, dove può portare. L'arte alla fine è solo un pretesto; quello che conta sono gli uomini, la vita degli uomini. Eppure, l'arte può avere una funzione politica, perché si occupa dell'uomo e della sua maniera di vivere: l'uomo che possiede anima e sentimento e fame di bellezza e di giustizia, che ha bisogno di conforto e di stimolo. Tutto ciò lo aveva capito duecento anni fa una donna: la duchessa Maria Luigia d'Austria, e questo edificio, questo Teatro, è un po' il simbolo del vasto progetto culturale di riforme che ella intraprese durante il suo Governo e che ha reso Parma più bella, più vivace, più ricca, permeandola della sua personalità e delle sue inclinazioni: l'arte, la musica, il buon cibo. si impegnò a ricercare la bellezza in ogni angolo, anche quello più sperduto e abbandonato, lavorando per realizzare progetti che potessero far ritrovare quella dimensione umana che, di solito, nel processo di una città, anche oggi va perduta. Non solo realizzò le più importanti opere pubbliche ancora funzionanti - il ponte allora più lungo d'Europa, i cimiteri - ma realizzò opere soprattutto a beneficio dei poveri. Anche in questo Teatro impose la vendita dei biglietti a prezzi ridotti per far entrare tutti i cittadini, anche quelli più svantaggiati. Pensò alle donne, ai malati di mente, fece allestire in un convento cittadino una struttura che è nota come l'Ospizio dei pazzerelli. Ieri abbiamo festeggiato le donne, richiamando i successi ottenuti anche di recente in questo ambito e oggi non possiamo, in questa occasione, non ricordare una donna che riuscì a precorrere i tempi in un mondo dominato dallo strapotere maschile. Si dedicò con particolare interesse alla condizione femminile, inaugurando l'istituto di maternità e la clinica ostetrica universitaria. Era una donna straordinaria che non amava il potere, non era ambiziosa, era di carattere gioviale, non era una rivoluzionaria, ma il suo Governo fu rivoluzionario. Nel Ducato fu donna e sovrana culturalmente illuminata. Maria Luigia ci insegna che la cultura della bellezza si può quindi estendere anche alla politica, all'economia e allo sviluppo di un territorio. Un Paese che non è governato da *leader* sognatori con una grande visione politica è un Paese senza futuro. Tecnici e burocrati non possono rendere grande una Nazione. La cultura è ciò che permette all'uomo di mantenere la propria dignità e la propria umanità. Il bello della cultura e la sua essenza profonda stanno nella gratuità, nella consapevolezza che in questo nostro mondo ingiusto ognuno deve fare la sua parte, rischiare, avere idee, inventare. Solo così, attraverso la fantasia e la creatività, possiamo immaginarci un mondo migliore. È per queste ragioni che il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questa proposta. comincio col dire che chiaramente il Gruppo del MoVimento 5 Stelle è a favore di questo provvedimento, lo è stato in Commissione, è stato a favore della procedura abbreviata la settimana scorsa

il Teatro Cilea di Reggio Calabria, (*Applausi*) il Teatro Rendano di Cosenza, il Teatro del Maggio musicale fiorentino, il Teatro Verdi di Firenze, il Teatro di Trieste, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Municipale di Piacenza, dove ha sede l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata e diretta dal maestro Riccardo Muti, i teatri cosiddetti di tradizione, che sono pezzi fondamentali della nostra storia e della nostra cultura e che sono pezzi di architettura e di ingegneria straordinari, che ci invidia tutto il mondo, come il Teatro Grande di Brescia

vi invito veramente ad andare a visitare. Credo che abbiamo l'obbligo, in quest'Aula, di considerare tutti i teatri, anche quelli di provincia, anche quelli meno importanti, che però sono un luogo di aggregazione fondamentale per tutti i nostri territori. Dobbiamo considerarli tutti

assistito al concerto di una formazione orchestrale proveniente dal Conservatorio di Trieste, rispetto alla quale noi tutti ci siamo alzati in piedi tre volte. Ecco, anche quello non deve essere un gesto di autoassoluzione rispetto a quello che possiamo fare. Ricordo infatti che le studentesse che abbiamo visto ieri fuori di qua non hanno futuro, non hanno un lavoro nel nostro Paese. Non possiamo semplicemente alzarci durante il loro concerto per riconoscere giustamente il loro valore artistico, ma dobbiamo dire a quelle ragazze e a quei ragazzi che nel nostro Paese passano dieci anni in conservatorio a studiare, che quando hanno finito di studiare c'è anche un lavoro, con dei contratti a tempo indeterminato e non a tempo determinato e sottopagati. *Commenti)*. No, è allucinante quello che non fate voi per la cultura da trent'anni in questo Paese, caro presidente Romeo, quello è allucinante. Detto questo, io credo che si debbano fare delle cose e in questa direzione vorrei ricordare che abbiamo depositato due disegni di legge con il MoVimento 5 Stelle che vanno nella direzione di essere propositivi. Il primo è quello che concerne gli asili musicali. Se vogliamo infatti che i giovani

legge, presentato in Commissione cultura, è volto a ripristinare i corpi di danza stabili all'interno delle fondazioni liriche. Anche al Teatro Regio di Parma si sono esibiti grandissimi ballerini di fama

che quello che stiamo facendo è una cosa giusta, è giusto invitare in quest'Aula delle formazioni orchestrali del nostro Paese, ma è anche giusto, una volta votato questo documento, far sì che gli investimenti per tutto il comparto culturale diventino più importanti di quelli che ci sono oggi.

che ringrazio per aver portato in Assemblea una discussione importante al fine di riconoscere monumento nazionale il Teatro Regio di una città, come quella di Parma che, grazie direttamente a Maria Luigia d'Austria, ha conosciuto lo sviluppo della cultura, della musica e dei valori della tradizione della musica italiana. È sicuramente importante riconoscere questo Teatro come monumento nazionale. Concordo con alcuni colleghi che hanno detto che mancano i fondi perché poi dichiararlo monumento nazionale Successivamente, nel caso in cui ci saranno problematiche e si vorrà direttamente investire sull'arte e sulla cultura, i fondi si troveranno. È giusto poi anche riconoscere altri monumenti nazionali

Però io dico a questi colleghi: nella scorsa legislatura, per cinque anni, siete stati in maggioranza. Cosa avete fatto? Invece di fare polemica in Aula, durante una dichiarazione di voto, ritengo importante farla in Commissione, con il Governo, per arrivare a delle proposte concrete e per portare avanti insieme le competenze per valorizzare questo settore. Mi rivolgo direttamente al sottosegretario Sgarbi, qui presente, che è venuto a visitare le terre verdiane. Questo è un anno importante e il Teatro Regio di Parma deve sicuramente essere incluso nella rete per la valorizzazione dei festeggiamenti per Verdi, come tutte le realtà del territorio del Granducato di Parma e Piacenza, perché sia il Teatro Regio che altre realtà possono raccontare la storia del maestro Verdi. Noi del Gruppo Lega, siamo i fautori di questa proposta di legge e riteniamo importante dichiarare il Teatro Regio di Parma monumento nazionale. Il nostro voto sarà sicuramente favorevole, come sarà favorevole, naturalmente, su qualsiasi altra proposta volta alla valorizzazione dell'arte e della cultura italiana sia a livello nazionale che nel mondo. *(Applausi)*.

colleghe e colleghi, Governo, mi fa molto piacere intervenire nuovamente su questa proposta, che condivido molto e che ci vede uniti nel giudizio di merito. Anche questo io credo rappresenti un po' la grande forza della cultura,

la stessa che ha accompagnato e che accompagna il Teatro Regio di Parma e che ci porta a dire qui oggi convintamente sì alla proposta di inserirlo tra i monumenti nazionali. La dichiarazione di monumento nazionale è doverosa per dare il giusto riconoscimento a un teatro come quello di Parma, considerato tra i più prestigiosi e noti al mondo. Fu inaugurato il 16 maggio del 1829, con «Zaira», un'opera che fu appositamente composta per l'occasione da Vincenzo Bellini. La sua costruzione, voluta - come hanno detto i colleghi - della duchessa Maria Luigia d'Austria, fu affidata all'architetto Nicola Bettoli; dopo otto anni di lavoro venne fuori un'opera imponente, un edificio di gusto neoclassico che oggi conta circa 1.200 posti a sedere. Il Teatro Regio di Parma, inoltre, contiene uno degli esempi più antichi e meglio conservati di camera acustica decorata, dipinta a tempera da Carmignani e composta da pannelli di canapa di forme e dimensioni diverse, da poco restaurati, con motivi che ripropongono la decorazione dei palchi della sala. Quando, Presidente, la settimana scorsa sono intervenuta sulla richiesta di procedura abbreviata *(Brusio)* - sento un mormorio ho fatto riferimento all'importanza della cultura in un tempo nel quale la guerra e la violenza soffiano prepotentemente e insistentemente alle porte dell'Europa. Vorrei ribadire un concetto che forse può aiutarci a comprendere quanto simbolico e quindi importante sia il provvedimento che oggi stiamo approvando. Abbiamo tutti, io credo, ben presente la furia dell'ISIS, intenta a distruggere monumenti e opere d'arte; allo stesso tempo mi ha colpito, invece, la generosità delle donne e degli uomini che, alla vigilia dei bombardamenti, hanno cercato con forza non solo di mettere in sicurezza se stessi, ma anche i materiali dei principali monumenti delle maggiori città ucraine. ucraine. Sono gesti che hanno un valore simbolico enorme. I primi sanno che con quella azione feriscono e cancellano la storia di un popolo; distruggendo i loro monumenti, infatti, distruggono una parte della loro cultura e della loro stessa identità. I colleghi sono molto interessati. I secondi, invece, sentono il bisogno di difendere quei monumenti che, al pari dei nostri, rappresentano appunto la loro storia, che è poi la storia di una comunità e di un Paese. Difenderli significa prendersene cura e valorizzarli. Significa dare dignità alla memoria che esse portano in sé. *(Applausi)*. Una memoria fatta di cultura; cultura che è libertà di pensiero, di espressione e, nel caso del teatro di Parma, cultura che è storia vivente. L'ho già detto, ma voglio ribadirlo ancora. Mi piace pensare alla cultura e alla conoscenza, in questo preciso momento storico, come ad un fenomeno che unisce i popoli nella pace, che sa riconoscere le persone. In un tempo di guerra come quello che stiamo vivendo in zone così prossime a noi la cultura e la musica sono il rifugio da ricercare per promuovere la pace. In particolare, i teatri sono luoghi sparsi in cui si coltiva l'umanità di un popolo, si radica la identità di una comunità, si insegna a guardare e riconoscere la bellezza: il teatro come bene comune. Naturalmente, bisogna sempre pensare a dare centralità alla cultura e alla conoscenza e, quindi, risorse e riconoscimento a tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo della cultura e dello spettacolo. Tanti sono gli attori teatrali del cinema che ci chiedono che il teatro e il cinema si insegnino a scuola. Non posso dimenticare le belle parole di un bravissimo attore, Pierfrancesco Favino, quando ci ha detto che le lezioni di teatro e cinema nelle scuole favoriscono la conoscenza. Dal teatro e dal cinema si impara tanta vita. Favorire conoscenza significa affollare i teatri; significa portare i giovani a stare insieme e a parlarsi; significa unire generazioni. Ancora, il cinema e il teatro che entrano anche nei luoghi di detenzione e nelle carceri minorili, diventando una finestra sul mondo, mondo, hanno la forza di salvare i giovani, di insegnare loro a vivere. Ce lo insegna in questi giorni il grande successo di una *fiction* come «Mare fuori», prodotta anche grazie al lavoro del servizio pubblico Rai. Rai. Signor Presidente, voglio inoltre ricordare la particolarità dell'orologio del Teatro Regio, che dal 1829 scandisce il tempo di opere e concerti e che, grazie a un lungo restauro, nel 2018 è tornato a funzionare. Quell'orologio è certamente il simbolo del tempo che passa, ma è anche, allo stesso tempo, un punto di riferimento per coloro che vivono quel teatro, che amano l'arte, la musica e quei luoghi meravigliosi che sono i nostri teatri. Mi piace pensare che oggi noi qui, tutti insieme, stiamo facendo la nostra parte.

di rappresentare la nostra Italia, la nostra arte, la nostra storia, la nostra cultura e la nostra tradizione. Grazie anche al relatore, che ci ha dato un po' la geografia del teatro. Per questo, signor Presidente, a nome del Partito Democratico, comunico che noi ci siamo e che, con il nostro voto favorevole, immaginiamo di scrivere un altro piccolo pezzo della grande storia della nostra bella Italia. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, sono lieto di intervenire per confermare il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo disegno di legge, che ereditiamo dalla precedente legislatura e quindi da un Parlamento differente e da un Governo differente. Ciò rende l'approvazione di questo disegno di legge oggi una cosa assolutamente non scontata, anche perché abbiamo avuto la capacità politica di adottare la procedura abbreviata, il che fa di questo provvedimento un atto approvato con

valorizza l'opera di una grande e illuminata donna del passato, la quale ci ha tramandato, grazie alla sua illuminata attività, l'eredità dell'atto che oggi approviamo. Maria Luigia ad Austria, come hanno già detto altri colleghi prima di me, era una sovrana culturalmente illuminata, che ha fortemente inciso sull'identità culturale di Parma, rimanendo nel cuore dei cittadini, avendo una eredità, non solo fisica, come patrimonio culturale, ma anche di grande valore per la comunità locale. Grande donna, per fortuna non unica. Infatti, mi viene da raffrontarla e paragonarla ad un'altra figura illustre del secolo precedente, che mi è più vicina, essendo fiorentina. Un'altra sovrana illustre, non comprimaria di sovrani che regnavano nel Settecento e nell'Ottocento. Parlo, in particolare, di di Anna Maria Luisa de' Medici, che, analogamente a Maria Luigia d'Austria, ha lasciato un patrimonio

con grande generosità e lungimiranza, ha saputo lasciare al popolo fiorentino all'epoca, ma, se guardiamo all'identità culturale nazionale, anche al mondo odierno.

loro operato politico nell'Italia dell'epoca. Tuttavia, sono lieto anche perché questo è un atto che sostanzialmente è l'applicazione pratica dei

che difendiamo un teatro che ha un valore storico, ma noi difendiamo soprattutto una identità culturale, tradizioni ed eccellenza, che sono elementi distintivi delle comunità. noi ci pregiamo di attuare una salvaguardia, senza arretrare, senza aver paura di apparire rivolti al passato, senza cedere a quel pensiero debole di chi vuol cancellare la cultura e le nostre radici.

Certo, essere conservatori non significa rimanere solo nel passato, ma conservare quel passato per garantire un futuro migliore. Noi scacciamo l'idea che il conservatore sia un uomo del passato, anzi è l'uomo del futuro, come del resto si può verificare anche dalle nostre prime iniziative di Governo. Io vorrei sottolineare le prime iniziative del ministro Sangiuliano su un tema che si coniuga con quello del Teatro Regio di Parma, proprio mettendo in sicurezza il patrimonio artistico non solo di Villa Verdi, ma anche il suo contenuto, quindi le opere che il grande compositore Verdi, a pochi chilometri da Parma, cioè a Busseto, ha saputo realizzare.

la polemica che si è letta sui giornali sia sopita. Mi risulta anche che, per fortuna, i gestori del Teatro Regio di Parma abbiano acconsentito a seguire le iniziative individuate per la valorizzazione di Villa Verdi, con tutte le iniziative a sostegno dell'acquisto della stessa e che sono diffuse in tutti i teatri lirici italiani. Per fortuna ci si sta rimettendo sui binari giusti, perché crediamo che il Teatro Regio di Parma debba avere un ruolo fondamentale nella valorizzazione dell'opera e della figura di Verdi e ribadisco e ribadisco che quello è il luogo più adatto rispetto ad altri. Come dicevo, però, chi opera nel solco dei conservatori non è solo custode delle tradizioni. Noi siamo consapevoli, come diceva qualche collega, del fatto che questo sia un atto quasi solo simbolico, quindi non possiamo accontentarci. Questo non può per noi essere un punto di arrivo, ma semmai un punto di partenza. Dico questo perché, come dicevano i colleghi, il provvedimento in esame non consente di fare un finanziamento pubblico a un monumento, seppur riconosciuto oggi come monumento nazionale. C'è quindi una necessità di valorizzare i beni culturali e questo lo si può fare solo affidandosi a soggetti gestori capaci di generare offerte culturali all'altezza e iniziative che rilancino il Teatro non solo come mero monumento e come luogo della memoria, ma anzi come luogo vivo e animato, come luogo di confronto, di dibattito locale e sociale, e dove manifestazioni di bellezza, arte, cultura e spettacolo

luogo di una grande tradizione operistica italiana. Lo dicevo prima: sarebbe bello rivedere anche qualche opera di Verdi rappresentata a Parma. Concludo sottolineando che oggi è l'inizio di un percorso. Auspichiamo che la valorizzazione trasformi questo monumento nazionale in un volano per la ripresa economica del Teatro: mi riferisco al fatto di saper attrarre visitatori quando non ci sono rappresentazioni (perché un monumento si va a visitare), ma saper anche raccogliere spettatori, cioè chi paga un biglietto per vedere uno spettacolo di alta qualità. Le risorse sono necessarie e credo che sia illusorio pensare - ne abbiamo parlato qualche volta anche in Commissione con il collega Pirondini con il collega Pirondini - che la cultura italiana e i nostri grandi teatri possano basarsi solo su risorse pubbliche. Ci auguriamo quindi che il principio della raccolta, tramite iniziative culturali, di risorse private abbia, invece

oggettivamente è illusorio pensare che solo con risorse pubbliche si possa garantire un'offerta culturale all'altezza in tutto il territorio nazionale. la sfida per i gestori del Teatro Regio è lanciata. Adesso sta a loro dimostrare che, con una grande offerta culturale, il Teatro può essere rilanciato. Il Governo sta facendo la propria parte. Ci auguriamo che il Teatro Regio faccia parte di quelle iniziative anche dal ministro Sangiuliano e che questo sia l'avvio di una grande stagione di rilancio non solo del Teatro come monumento, ma come offerta culturale.

è con compiacimento e stupore che prendo atto del voto favorevole all'unanimità e per alzata di mano, che non vedevo, a memoria di una lunga esperienza parlamentare (benché più breve di quella del senatore Casini), da quando in quest'Aula da quando in quest'Aula vidi votare i democristiani, dopo un voto ambiguo della Commissione che aveva esaminato il caso del processo Andreotti, all'unanimità contro il senatore Andreotti per mandarlo a processo: una pagina triste della storia italiana. Si votò per alzata di mano. Quindi rivederla di colpo è come tornare indietro di trent'anni, rispetto a procedure che il Parlamento non applica, e mi dà il senso anche di un'acclamazione, di una volontà che nel caso di Andreotti era di giustizia, sia pure negata alla verità, e oggi è di una giustizia nei confronti della cultura, che avete evocato in modo così unanime e perfino in modo polemico. benché le osservazioni della senatrice Murelli, che è la proponente del disegno di legge, in questo momento siano abbastanza corrette, nel senso che non c'è colpa. Semmai, c'è colpa per tutti, per non aver fatto quello che ha detto in modo in modo molto preciso il senatore Pirondini, che è un uomo dotto e colto, nonostante la sua presenza in banchi che sono adusi a polemiche talvolta strumentali. Ma in questo caso ha detto una cosa perfetta, e cioè: perché soltanto il Teatro Regio di Parma? Ogni teatro è monumento nazionale: un monumento nazionale dell'arte, della musica, della storia, della memoria. Faccio fatica a immaginare che non lo sia il Teatro San Carlo di Napoli. Qui avete scritto una di quelle formulette che, in un disimpegno sostanziale e forse sbagliato, recita: recita: determinare la neutralità finanziaria. Come se la neutralità fosse una questione di guerra. Neutralità vuol dire «non vi diamo soldi» o che non ci sono soldi, che è cosa comunque sbagliata rispetto alla cultura. Questa neutralità vuol dire nella sostanza che non costa nulla

il pregevole orologio che scandisce il tempo. Ogni orologio scandisce il tempo e non è che sia pregevole in quanto è un riferimento decorativo o artistico. Quindi è stato evocato perché più si perde tempo nello stabilire che i teatri sono monumenti nazionali, più si perde

nella precedente legislatura e che, come singolarmente accade, visto il procedere dal Governo verso il Parlamento, è di iniziativa parlamentare. Questa cosa mi pare la più bella di tutte, ovvero che sia

consapevolezza e il compiacimento del fatto che Parma è molto importante, perché è la città di Verdi. Non dimentichiamo però che, se qui non abbiamo oneri o abbiamo neutralità finanziaria, per Puccini, il cui valore è pari a quello di Verdi, è stato stanziato un finanziamento intorno ai 9 milioni di euro per il *festival* e l'attività di un luogo, sta avvenendo - lo dico a tutti i parlamentari: oggi vedrò il sindaco di Viareggio - la distruzione del piazzale davanti alla villa, che il sindaco ha ritenuto di di cambiare, buttando giù i pilastrini, che sono importanti non meno del citato orologio. Quindi esorto tutti voi a vigilare anche sul fatto che poi, nel nome delle celebrazioni, non si dimentichino la storia e la memoria di un luogo, che come i luoghi di Gozzano, è un luogo della poesia, delle cose povere, delle cose piccole, di piccole aiuole. Comunque oggi cercherò di spiegare al sindaco di Viareggio che si può onorare Puccini anche senza fare una pista per gli elicotteri davanti a casa sua. Detto questo, colgo appunto l'occasione per segnalare l'opportunità di ascoltare le parole del senatore Pirondini in merito ai monumenti nazionali, che ha elencato e cioè quei teatri in cui si celebra per tutti, per l'Italia e per il mondo, la grandezza della musica, nel nome dei valori che avete ricordato, della pace e della neutralità, in questo caso rispetto alla divisione ideologica, perché la musica unisce tutti, destra e sinistra. Se unisce tutti, ogni teatro è monumento nazionale, per cui si cominci da Parma e si proceda per tutti i grandi teatri italiani.

finestra") sui ritardi nell'erogazione dell'assegno unico e universale da parte dell'Inps.

sociali*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Murelli per aver portato all'attenzione del Governo la questione avente ad oggetto le misure che si intendono adottare, al fine di garantire l'accredito puntuale da parte dell'INPS dell'assegno unico familiare. Questo Governo, nella legge di bilancio approvata di recente, ha disposto un cospicuo aumento delle somme stanziate per l'assegno unico e universale quale beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari per il periodo proprio che va dal marzo di ciascun anno a febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente. La misura, infatti, è stata rafforzata dal Governo proprio per aiutare le famiglie numerose e dare maggiore sostegno alle persone con disabilità, alle persone di minore età con disabilità. Dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50 per cento dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e, per i figli con un'età compresa da uno a tre anni, per le famiglie con tre e più figli con ISEE fino a 40.000 euro. È prevista anche una maggiorazione del 50 per cento dell'assegno unico per le famiglie con quattro o più figli. Sono confermate e rese e strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Con riferimento alla problematica segnalata, si rappresenta che si è provveduto a condurre un'approfondita istruttoria, volta ad acquisire utili elementi da parte dell'Istituto di previdenza, al fine di dare una compiuta ed esaustiva risposta. A tale proposito, l'INPS ha dichiarato che i pagamenti sono eseguiti tramite Banca d'Italia e ammontano a circa 1,3 miliardi di euro al mese, corrispondenti a oltre 5,5 milioni di bonifici mensili. Nella prima decade di ogni mese l'Istituto provvede a istruire le domande di assegno unico nonché a svolgere tutte le eventuali lavorazioni di carattere straordinario come, ad esempio, arretrati e conguagli. Terminate le istruttorie, l'INPS trasmette i mandati di pagamento alla Banca d'Italia, che procede ai relativi versamenti nel limite massimo stabilito di circa 4 milioni di bonifici per data regolamento, e cioè il giorno in cui una transizione o contratto devono essere regolati e contabilizzati. Le date di regolamento dei bonifici dei bonifici per la regolazione dell'assegno unico sono state concordate tra il 12 e il 20 del relativo mese di competenza ed eventuali accrediti non eseguiti in tale arco temporale vengono inseriti nel flusso ordinario di erogazione delle altre prestazioni di competenza dell'Istituto. Per ciò che concerne la segnalazione dei ritardi nell'erogazione dell'assegno unico, l'INPS ha precisato che, dalle verifiche operate sui flussi di pagamento del 2022, è emerso che i rallentamenti si sono verificati esclusivamente nei primi mesi di avvio dell'attività. L'INPS ha altresì dichiarato che, nel solo mese di settembre 2022, a fronte del volume eccezionale di prestazioni effettuate, sono stati riscontrati disservizi per circa 600.000 bonifici, pari a 142 milioni di euro, e corrispondenti all'11 per cento circa delle erogazioni mensili. L'Istituto ha precisato che, in questa eccezionale occasione, l'erogazione è stata posticipata di non più di cinque giorni lavorativi (questo è ciò che ha sottolineato l'Istituto). Più in generale, secondo quanto riferito dall'INPS, non può parlarsi propriamente di ritardi nei pagamenti della prestazione dell'assegno quanto piuttosto della non predisposizione di date fisse mensili, nelle quali gli stessi pagamenti sono accreditati agli utenti. Infatti, i pagamenti avvengono con regolarità ogni mese sin dall'avvio della prestazione, mentre le date di effettiva disponibilità delle somme da parte dei beneficiari finali possono arrivare da un mese all'altro e variare. Nell'evidenziare l'importanza della questione sollevata, si rassicura la senatrice interrogante che l'INPS si sta adoperando con il massimo impegno per svolgere tutti gli approfondimenti volti a garantire le modifiche gestionali e le implementazioni informatiche per assicurare che il pagamento avvenga con cadenza stabile. La soluzione auspicata è quella di rimodulare la tempistica della procedura dei controlli sulla presenza dei requisiti di legge per beneficiare dell'assegno unico e universale al fine di consentire la calendarizzazione degli accrediti in un ristretto numero di date valuta prefissate. Concludo sottolineando che sarà cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilare sull'attuazione da parte dell'INPS delle modifiche gestionali, nella piena consapevolezza che l'assegno unico rappresenta un'importante misura di sostegno economico per i nuclei familiari e per tale motivo è certamente priorità di questo Governo attenzionare questa misura e la capacità dell'INPS di essere efficiente, efficace e tempestivo senza che nessuna famiglia

perché questa è l'attenzione che il Governo deve avere rispetto alle famiglie. Non ci possono essere ritardi o problemi nelle procedure di erogazione dell'assegno unico, perché in precedenza l'assegno per i figli veniva versato e pagato direttamente regolarmente

per sostenere la famiglia e per sostenere la natalità nel nostro Paese.

Dopo anni di assenza, lo scorso 8 febbraio ho partecipato, con il vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Fruit Logistica 2023 di Berlino, la più grande fiera professionale al mondo del settore ortofrutta. La presenza del vice ministro Cirielli è stata fortemente voluta dal presidente Meloni per simboleggiare quanto il nostro agroalimentare sia un elemento centrale che ha l'Italia per presentarsi all'estero. In tale contesto, è emersa l'estrema necessità di promuovere politiche che diano risposte concrete ad un settore che soffre per il calo dei consumi interni, il notevole aumento dei costi, le condizioni climatiche disastrose, i fitopatogeni aggressivi e lo scarso riconoscimento di un settore che è trainante non solo per l'agricoltura italiana, ma anche per l'economia stessa del Paese, a partire dal suo cruciale ruolo occupazionale in molte Regioni. Detto questo, rilevo che riguardo alle iniziative per compensare la perdita di liquidità delle imprese del comparto, nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM), disciplinata dai regolamenti UE/1308 e UE/2021, sono presenti molteplici interventi in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli anche di carattere finanziario. Infatti, la vigente normativa unionale e nazionale di riferimento prevede il finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute attraverso un aiuto comunitario generalmente pari al 50 per cento delle spese incluse in alcuni specifici programmi di attività, definiti programmi operativi. All'interno dei predetti programmi trovano spazio interventi dedicati agli investimenti, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle condizioni di commercializzazione, all'ottimizzazione dei costi di produzione, nonché alla prevenzione della crisi e gestione dei rischi. In particolare, in relazione al 2023, le organizzazioni di produttori del settore hanno presentato alle competenti Regioni 256 programmi operativi, approvati per un aiuto unionale complessivo pari a circa 300 milioni di euro annui.

con un contributo fino al 70 per cento della spesa premi, sostenuto dagli agricoltori, a copertura dei rischi da avversità atmosferiche, tra cui anche la siccità. Occorre poi considerare che per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva l'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha esteso anche alle imprese agricole che non hanno stipulato la copertura assicurativa per i danni da siccità subiti dal maggio 2022, la possibilità di accedere agli interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. La norma reca una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro. Attualmente, le Regioni stanno raccogliendo le domande da parte dei beneficiari e, sulla base dei fabbisogni che verranno comunicati in esito all'istruttoria, si procederà alla ripartizione delle somme tra le Regioni. Segnalo inoltre che a partire da quest'anno, nell'ambito del piano strategico nazionale, è prevista l'attivazione di un nuovo strumento di intervento *ex ante* finanziato con le risorse dell'Unione europea sotto forma di fondo di mutualizzazione nazionale, cui potranno accedere tutte le imprese agricole per fronteggiare i danni a carico delle colture in caso di eventi catastrofali quali la siccità ed ottenere così un ristoro in tempi compatibili con le esigenze finanziarie aziendali per garantire la pronta ripresa economica e produttiva. La novità dell'intervento risiede nel fatto che sarà costituito esclusivamente da risorse comunitarie senza alcun esborso per gli agricoltori, grazie alla possibilità di finanziare con le risorse del primo pilastro della Politica agricola comune (PAC) la quota del 30 per cento a carico dell'agricoltore, coprendo il restante 70 Fondo europeo di sviluppo regionale. Riguardo poi alle misure volte a rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, ricordo che la legge di bilancio 2023, al fine di incentivare la ripartizione economica del tessuto imprenditoriale del Paese, ha istituito nello stato di previsione del Ministero il Fondo per la stabilità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Anche per il settore in esame il Fondo ha l'obiettivo di ridurre i costi sostenuti per la produzione delle imprese agricole, sostenere le relative filiere e gestire la crisi di mercato. Al fine di rendere costante e puntuale lo scambio di informazioni sull'organizzazione di mercato tra le diverse componenti interessate e di gestire le eventuali situazioni di crisi, è nostra intenzione implementare le attività del tavolo frutticolo nazionale, già istituito con decreto del 6 marzo 2020. Infatti, proprio ieri, con il ministro Lollobrigida abbiamo incontrato i maggiori rappresentanti del settore ortofrutticolo, affrontando alcuni dei principali temi che preoccupano il comparto, quali il prezzo equo, l'*import-export*, la produttività della filiera, la siccità e gli imballaggi. È stata un'importante occasione di aggiornamento e di confronto per ascoltare le istanze dei protagonisti del comparto ed elaborare insieme, ragionando come sistema Italia, soluzioni e prospettive di sviluppo per un settore fondamentale del *made in Italy*. Il nostro compito è sostenere questo comparto attraverso un piano di rilancio del settore, non solo per affrontare le emergenze, ma anche per assicurare uno sviluppo solido e sostenibile. Puntiamo con forza sulla sinergia con altri Ministeri, come confermano i tavoli con i Dicasteri di salute, lavoro e *made in Italy*. In questo modo il sistema Italia può essere ancora più competitivo. di un primo passo al quale seguiranno specifici incontri per risolvere le problematiche del comparto anche in un'ottica strategica che garantisca alle nostre produzioni di qualità di essere ulteriormente valorizzate in termini promozionali e conquistare nuove fette di mercato in Italia e all'estero.

presenti sono piemontesi come me e li saluto volentieri. signor Sottosegretario, per la risposta. Io credo che dentro ci siano alcuni passaggi importanti, come il sostegno alla produzione e all'*export* e quello che è stato fatto.

In Piemonte (sono partito dai dati del nostro territorio) abbiamo 8.000 aziende impegnate nel settore, su quasi 19.000 ettari, ma le problematiche vere che sta vivendo la prima parte della filiera sono costituite da una carenza enorme di liquidità,

legislatura), a gestire questa fase e ad aprire a questa possibilità di rimodulare i mutui a venticinque anni, con due anni di preammortamento, magari inserendo anche una condizione di tasso che non sia da strozzinaggio, fatto che diventa fondamentale.

all'ora. Credo che questi temi debbano essere affrontati insieme a quelli grandi, come i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché è la quotidianità che rischia di far chiudere le nostre imprese e le nostre aziende agricole. Tenga presente che il discorso di avere un onere contributivo inferiore riguarda 120.000 imprese nel nostro Paese, ma i lavoratori in agricoltura sono 1,05

Non possiamo più permetterci che i contadini e gli agricoltori italiani lavorino senza la garanzia di un ricavo. *(Applausi)*. E lei lo sa bene, perché lo sosteneva con me nella scorsa legislatura ed eravamo d'accordo su questo tema. La ringrazio pertanto per il contributo che ha dato, soprattutto come risposta, a tutti coloro che oggi la stavano attendendo. Dall'altra parte, le chiedo ancora uno sforzo. Noi contribuiamo come Commissione (il presidente De Carlo e i miei colleghi tutti) per far sì che si possa veramente arrivare a una soluzione ottimale di questo problema e il settore ortofrutticolo possa essere finalmente risollevato.

Signor Presidente, in relazione al grave evento citato, accaduto nella notte tra il 7 e l'8 agosto 2022, si evidenzia che in quel periodo presso l'Istituto era stata raggiunta la capienza massima, anche a causa delle necessarie misure precauzionali adottate per limitare i rischi di infezione da Covid-19, in ragione delle quali occorreva garantire, nella fase di accoglienza, la disponibilità di stanze che consentissero l'isolamento precauzionale, come previsto dalla vigente circolare del Ministero della salute. Ciò premesso, risulta che il minorenne era stato temporaneamente allocato presso una stanza del locale infermeria, naturalmente previa compiuta valutazione effettuata dall'*équipe* dell'istituto, in considerazione delle difficoltà di inserimento nel contesto detentivo, dovute al fatto che il ragazzo sperimentava il suo primo ingresso in un istituto penale minorile. Il 6 agosto 2022, in ragione della sopravvenuta inagibilità del reparto infermeria, dovuta al danneggiamento dei locali conseguente ad un evento critico di cui si rendeva responsabile un altro minorenne, veniva effettuato lo spostamento del giovane dal locale infermeria a una stanza di diverso reparto, che era occupata anche da altri ragazzi e che rappresentava, in quel frangente, l'unico posto detentivo disponibile. Purtroppo, nella notte tra il 7 e l'8 agosto, per come riferito per come riferito dal giovane, venivano perpetrate violenze a suo danno da parte dei suoi compagni di cella, due minorenni e un giovane adulto di diciott'anni. La mattina dell'8 agosto, il minorenne, a seguito del colloquio con l'educatore, dove raccontava le violenze subite, veniva nuovamente trasferito nel reparto infermeria, dove nel frattempo si era resa disponibile una stanza, a seguito del ricovero del giovane che aveva messo in atto i danneggiamenti sopramenzionati. Acquisite tali informazioni, il giovane veniva altresì immediatamente visitato dal medico dell'istituto e, su disposizione di questi, accompagnato, in data 9 agosto 2022, dapprima presso l'ospedale San Carlo di Milano e, successivamente, presso il Pronto soccorso violenza sessuale istituito presso la clinica Mangiagalli di Milano, e ciò per gli ulteriori approfondimenti specialistici. Si attivava inoltre l'immediato allertamento del personale dell'istituto, a seguito delle tensioni che inevitabilmente si erano venute a creare tra tutti i ragazzi al diffondersi della notizia di quanto accaduto, e si adottavano altresì provvedimenti per la salvaguardia del minorenne, attraverso la previsione di un regime di alta sorveglianza e il divieto di incontro con i ristretti nelle altre sezioni detentive, ciò principalmente al fine di scongiurare le criticità che potevano scaturire dalla diffusione della notizia tra i giovani detenuti. Contestualmente e doverosamente veniva inoltrata, al pubblico ministero di turno presso la competente procura della Repubblica, la *notitia* *criminis* nei confronti dei ragazzi indicati come autori delle violenze, dando corso altresì alle informative di rito al magistrato di sorveglianza e agli uffici superiori. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla giovane vittima nelle varie sedi in cui è stata ascoltata e visitata, il competente ufficio del Dipartimento ha effettuato il trasferimento in altri istituti dei due minorenni coinvolti negli abusi, mentre per il giovane adulto coinvolto si è provveduto a chiedere all'autorità giudiziaria competente il nulla osta al trasferimento presso una struttura detentiva per adulti, essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione del trattamento in ambito minorile,

ha riferito che pende procedimento penale a carico di due persone minorenni, peraltro entrambe detenute per altri fatti. riguardo risulta che, in data 27 dicembre 2022, è stata eseguita ordinanza custodiale in danno dei due indagati minorenni e che è stata richiesta l'audizione della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio. Venendo alle generali problematiche del sovraffollamento delle carceri e alle potenziali misure volte alla deflazione della nota criticità, mi pregio ribadire quanto già relazionato in risposta ad altre interrogazioni di pressoché analogo tenore.

nell'ambito delle disponibilità esistenti, di spazi immediatamente utilizzabili e, contemporaneamente, sono stati progettati nuovi istituti. Nel tempo, quindi da marzo 2014, sono stati istituiti ufficialmente l'applicativo spazi-detenuti il relativo gruppo di lavoro, con il quale sono state fornite ulteriori indicazioni riguardanti la locazione di spazi vitali minimi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e diventando, questo strumento informatico, allo stato il sistema più avanzato per definire l'insieme di relazioni tra detenuti e spazi detentivi. Tale applicazione consente non solo di conoscere il numero dei detenuti presenti nei singoli istituti, ma anche la loro corretta collocazione all'interno di ogni istituto, camere di pernottamento e lo spazio disponibile per ciascun individuo, consentendo così di verificare in tempo reale il rispetto dei parametri CEDU ed eventuali violazioni, con conseguente ripristino della legalità. Questo applicativo è peraltro utilizzabile dalla magistratura di sorveglianza, preposta per legge alla vigilanza sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) è costantemente ed anche attualmente impegnato in un programma teso all'aumento del numero dei posti detentivi mediante il recupero dell'agibilità di quelli indisponibili per carenze manutentive, nonché all'edificazione di nuovi padiglioni in penitenziari già attivi, come pure alla riconversione a uso detentivo di strutture demaniali dismesse, in particolare caserme, aventi caratteristiche tali da poterne prefigurare, prevalentemente con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, un possibile adattamento a istituto penitenziario. Tra il 2020 e i primi mesi del 2021 sono stati ultimati e attivati quattro nuovi padiglioni da 200 posti ciascuno presso gli istituti di Parma, Trani, Lecce e Taranto. Attualmente sono in fase di collaudo, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nuovo padiglione dal 92 posti destinato all'applicazione del regime previsto dall'articolo 41-*bis* presso la casa circondariale di Cagliari e il padiglione da 200 posti della casa di reclusione di Sulmona. Entro il 2023, inoltre, dovrebbe essere ultimato il padiglione da 200 posti che si sta realizzando presso la casa circondariale di Bologna, nonché quello da 400 posti in costruzione presso la casa circondariale Roma Rebibbia. Tra gli interventi avviati per il riadattamento e il riuso di strutture militari dismesse, si annota quello relativo alla caserma «Barbetti» di Grosseto, d'imminente presa in consegna da parte dell'amministrazione penitenziaria, da riconvertire in istituto da 400 posti. Inoltre, effettuati i relativi appalti dei lavori, entro il 2025 dovrebbero essere ultimati il nuovo padiglione da 200 posti presso la casa circondariale di Bologna e il nuovo istituto di Forlì, da 250 posti. Nell'ambito dei fondi complementari al PNRR, è stata prevista la realizzazione di otto padiglioni da 80 posti detentili, da edificarsi in aree già nella disponibilità di quest'amministrazione quali sedi di istituti di pena (Vigevano, Rovigo, Perugia, Viterbo, Civitavecchia, Santa Maria Capua Vetere, Ferrara e Reggio Calabria), con il duplice obiettivo sia di ampliare la recettività del sistema penitenziario nazionale, sia di favorire una permanenza nei luoghi di detenzione più dignitosa. Il *format* di questi padiglioni detentivi, di ispirazione fortemente trattamentale, è stato elaborato dalla commissione per l'architettura penitenziaria, costituita nel gennaio del 2021. La concreta attuazione di tali opere è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei con cui si è avviata un'opera di costante collaborazione finalizzata alla tempestiva attuazione dei progetti. La realizzazione di tali otto padiglioni dovrà essere ultimata entro l'anno 2026 e produrrà 640 posti detentivi. Ciò consentirà di contrastare con maggiore adeguatezza ed efficacia la problematica relativa alla condizione di sovraffollamento che affligge il sistema penitenziario, nonché di assicurare maggiore disponibilità di spazi utili al superamento dell'attuale criticità legata anche e soprattutto alla grave mancanza di superfici e ambienti e ambienti per le attività trattamentali. Infine, in ordine all'adozione di misure alternative al carcere, allo stato si evidenzia il recente intervento normativo di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, contenente appunto, tra le altre, la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Merita peraltro segnalare gli effetti e gli interventi nello specifico settore disposti con la legge n.

del Ministero della giustizia è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025. Tale Fondo è destinato a progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti detenuti mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università, nonché con i soggetti associativi progetti destinati all'assistenza ai detenuti; alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica; al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze; all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

di personale con posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Al comma 864 dell'articolo 1 si autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria sino al 2026 al 2026 (in diversi scaglioni). E ancora: all'articolo 6, comma 2, si autorizza la riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute SpA, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato. Concludo osservando che la risposta a questa interrogazione mi permette anche di segnalare un ulteriore elemento. Oltre al tema sollevato dall'interrogante

Se il sì è a utilizzare e a spingere sulla misura alternativa, il no è sicuramente per i provvedimenti che hanno il solo scopo di svuotare le carceri,

(che può intervenire nel nostro sistema carcerario), si possa incidere veramente nel recupero del soggetto. Questo va in favore del singolo, ma anche della nostra comunità, perché il soggetto che esce dal carcere, se ha imparato qualcosa,

hanno imparato qualcosa, si sono formati, sono stati rieducati e hanno aderito a un programma di rieducazione rientra nel circuito criminale. Credo che questo sia il vero investimento, al di là di quello sulle misure alternative, che già ci sono. Penso che su questo dobbiamo lavorare e massima è la nostra concentrazione, perché il beneficio è non solo per la singola persona, ma per tutta la nostra comunità.

tratta di un ragazzo che è stato fatto oggetto di violenza anche sessuale all'interno di una struttura dove in teoria bisognava pensare alla sua rieducazione e alla sua protezione. Tra l'altro, come succede di solito, e ancora di più vale per i minori, occorre chiedersi perché questo ragazzo fosse in prigione quello fosse il posto giusto. Aveva sicuramente commesso qualcosa di non giusto, di non etico e di antigiuridico, quindi probabilmente meritava anche una sanzione,

nel leggerle le avrà trovate evidentemente inaccettabili, considerando la tragedia che il ragazzo ha dovuto affrontare.

ha anche citato la legge di bilancio, con gli interventi che sono previsti, ma noi tutti ricordiamo che accanto alle assunzioni ci sono anche tagli sostanziali al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che non avremmo voluto vedere. Signor Sottosegretario, delle due l'una. O decidiamo di

non sono una realtà, ma abbiamo - giustamente - chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari, pertanto le persone con problemi psichiatrici sono ancora nelle carceri; sappiamo che l'anno scorso abbiamo avuto 84 suicidi, *record* di cui certamente non possiamo andare orgogliosi, ma che costituisce una macchia sulla nostra coscienza collettiva nazionale. Oppure, evidentemente, è importante che investiamo sulle carceri, che diamo una mano anche alla polizia penitenziaria e ai nostri direttori, che fanno

Bollate. Voglio dire dunque che abbiamo preso con grande serietà le parole dette dal ministro Nordio all'inizio di questa vostra esperienza di Governo su un uso più intelligente, più sensato - come diceva lei - e anche più egoisticamente logico del carcere: se le persone che escono non delinquono, è un interesse prima di tutto della società. Molto bene, ma vi aspettiamo sui fatti, signor Sottosegretario, perché vi ricordo sempre che il primo atto che avete adottato è stato introdurre un reato sui *rave*, con sei anni di reclusione, che servivano per consentire le intercettazioni. Dunque, il peggiore armamentario manettaro che si possa pensare è quello che ci avete fatto vedere nella pratica. Se alle parole del ministro Nordio, alle quali si aggiungono le sue, alate, di questa mattina, seguiranno i fatti, Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope ne saremo veramente molto lieti, per il bene del Paese. finestra") sulla gestione dei beni mobili e immobili sequestrati alla criminalità organizzata. dev'essere immediatamente posto in risalto che il Fondo unico giustizia è gestito dalla SpA Equitalia giustizia, la quale versa allo Stato le somme confiscate dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'utile della gestione finanziaria delle risorse liquide del Fondo unico giustizia e una quota delle risorse sequestrate stabilita con decreto ministeriale in base ai criteri statistici che tengono conto delle priorità e probabilità di restituzione. Dalla data di istituzione del fondo a oggi, le somme complessivamente riversate allo Stato consistono in circa 1,4 miliardi per provvedimenti giudiziari di confisca e devoluzione. Ciò è comprensivo di anticipazione di somme sequestrate e utile della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia dell'anno precedente. Le somme riversate allo Stato sono destinate alla riassegnazione in misura non inferiore a un terzo al Ministero dell'interno e in misura non inferiore a un terzo al Ministero della giustizia. Per il resto, entrano nel bilancio dello Stato. Le quote di riassegnazione sono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I DPCM finora emanati hanno sempre previsto la destinazione delle quote di riassegnazione nella misura del 49 per cento al Ministero dell'interno, 49 per cento al Ministero della Con specifico riferimento all'anno 2023, considerato che nel bilancio risulta già iscritta la somma di 30 milioni di euro sul capitolo 1537, a titolo di anticipazione della quota del fondo spettante a questo Dicastero per l'anno in corso, sono state invitate le articolazioni ministeriali a comunicare le esigenze riferite al finanziamento degli interventi tesi al funzionamento e potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, indicando i corrispondenti capitoli di bilancio sui quali allocare le risorse e il grado di priorità di ciascun intervento da sottoporre alla valutazione del Ministro. Per quanto attiene più specificamente alla destinazione a scopi sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, occorre ribadire che il decreto legislativo n. 159 del 2011, cosiddetto codice antimafia, agli articoli 45 e 49, stabilisce - con riferimento ai beni immobili definitivamente confiscati - un articolato sistema di prioritaria destinazione al patrimonio indisponibile dell'ente territoriale in cui il bene è situato. Il trasferimento al patrimonio indisponibile degli enti territoriali per la gestione finalizzata a scopi sociali non priva l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di stringenti poteri di verifica e di controllo. poteri di verifica e di controllo. Come si evince dal contesto dell'ultima relazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tale Agenzia ha proseguito la mappatura dei beni già consegnati, evidenziando le cause di mancato utilizzo e avviando tutte le azioni a sostegno dell'ente destinatario per una corretta ed effettiva utilizzazione. Può quindi sostenersi che l'attuale sistema di acquisizione e gestione delle risorse sequestrate e confiscate sia già orientato a consentire la loro destinazione all'utilità collettiva dell'ente territoriale soggiogato o comunque infiltrato dalla criminalità mafiosa, secondo le disposizioni richiamate. In ogni caso, segnalo che è allo studio di questo Dicastero l'introduzione di una modifica del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, volta a consentire il prelievo delle rilevanti giacenze del Fondo unico, quindi somme di denaro occorrenti ad affrontare, da un lato, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili confiscati destinati a usi sociali e, dall'altro lato, la promozione di attività sociali, a tal guisa restituendo, ai territori sottoposti al potere della criminalità organizzata di stampo mafioso, una porzione delle risorse alla stessa sottratte.

Sa cosa penso, signor Sottosegretario? Penso che sia stata una grande intuizione, perché certamente la mafia va combattuta sul piano della repressione criminale con le manette, con il carcere e bisogna essere il più efficaci possibili. Ma sappiamo anche che la criminalità organizzata vive anche di una sua coreografia, di un suo modo di imporre il proprio giogo sulle comunità nelle quali si infiltra, che è anche visibile.

E allora quando lo Stato decide ed è capace di sottrarre quegli strumenti, quelle insegne del potere di restituirle non soltanto ai territori che soffrono di quella violenza, ma di farli diventare momenti di rinascita civile, sociale e repubblicana, è lì che mostra la sua forza tranquilla,

E quindi la dobbiamo difendere, dobbiamo fare in modo che sia effettiva. Eppure, oggi ancora non lo è. Ci sono sicuramente delle bellissime esperienze. Non dimenticherò mai di aver visitato Radio Siani da Sottosegretario all'interno, una radio una radio fatta nel Comune di Ercolano di fronte al municipio dove i ragazzi nella casa del *boss* hanno creato una radio antimafia intitolandola a Giancarlo Siani, sul corso principale di Ercolano. È un dito in un occhio, ha veramente una potenza simbolica enorme, ma noi di queste esperienze dobbiamo averne sempre di più. Quello che succede è che spesso, però, purtroppo, quei beni arrivano alle associazioni anche dagli enti locali, magari dopo anni di incuria, magari perché vengono rovinati da chi non vuole che vengano riutilizzati. Dobbiamo fare in modo, allora, che l'assegnazione di quei beni non si risolva in un atto burocratico e formale, ma che lo Stato, oltre ad assegnare il bene, si preoccupi preoccupi di seguirne la rinascita, che metta chi va a gestirlo in condizioni di trasformarlo dal rudere che era in un luogo di vita civile. Per fare questo abbiamo bisogno di fondi. La stranezza di questo meccanismo è che i beni sequestrati e confiscati vengono poi allocati alle associazioni del terzo settore; i soldi che invece vengono confiscati al *boss* mafioso finiscono in questo Fondo unico per la giustizia. Quindi, il bene immobile prende una strada, i fondi ne prendono un'altra. Ma quei fondi dovremmo considerarli serventi rispetto allo scopo principale. Ho ascoltato con attenzione, e ne sono lieto, le sue parole. Vi seguiremo e vi sosterremo nella direzione, se vorrete prenderla, di riportare la vicenda su un piano più logico e dire che, quando c'è un sequestro di beni immobili e quei fondi in linea prioritaria vengano destinati al recupero di quei beni immobili che devono essere assegnati. Anche perché fa urlare al cielo per la rabbia l'idea che ci siano delle giacenze

di restituire visibilità alla democrazia e al vivere civile in tante nostre Regioni del Sud e - mi lasci dire - non soltanto del Sud, perché questi fenomeni - ahinoi sono sempre più diffusi anche nelle Regioni settentrionali del Paese. Proviamo a sistemare questa situazione, che sembra più un intoppo burocratico che altro, e a mettere questa bellissima legge, nata dalla grande idea di Pio La Torre, nelle condizioni di funzionare.

in data 21 febbraio, perché la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, dopo la sentenza del Ruby-*ter*, invece di prendere atto della sentenza, si è lasciata a commenti che io che io definirei politici. Un procuratore può fare le sue accuse, poi c'è il giudizio. Mi è sembrato che fossero attività improprie e per tale ragione ho sollecitato un'attività ispettiva. Lo stesso ho fatto il 23 febbraio

È francamente sconcertante questo perdurare di un'invadenza, in violazione del principio della separazione dei poteri - esecutivo, legislativo e giudiziario - che non posso immaginare

preoccupazione per la ritornata, rinnovata e reiterata invadenza della magistratura e addirittura l'intimidazione sull'attività ispettiva di un parlamentare. **Atti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

La seduta è tolta